Signor Presidente, oggi è il 13 dicembre 2006. Credo che non possiamo far passare questa data senza ricordare il colpo di Stato con il quale, il 13 dicembre 1981, il comunismo morente tentò di imporre ancora la propria regola totalitaria alla Polonia e a tutta l'Europa. Voglio ricordare in questo giorno le 30-40.000 persone che in una notte furono prese dalle loro famiglie, internate in campi di concentramento e delle quali si perse ogni notizia e contatto. Lei ricorderà, signor Presidente, anche la grande risposta del popolo italiano in quella occasione e il grande moto di solidarietà che sorse da gran parte di questo popolo. Voglio ricordare il ruolo che ebbe Comunione e Liberazione, il ruolo che ebbe la CISL con il suo personale impegno nella costituzione della Società degli amici della Polonia,

Voglio, in modo particolare, ricordare quella domenica. Ricordo - e anche lei forse ricorderà - l'atmosfera che si era creata: in Polonia si era alla vigilia dell'insurrezione. Ricordo di aver parlato alle Cappellette quella notte con Bohdan Cywinski, che lei conosce, che mi spiegava lucidamente: «Cosa faremo adesso? L'insurrezione è l'unica via. Impiccheremo tutti i comunisti, poi verrà l'Armata rossa e ci saranno un milione di morti». Quella domenica apparve Giovanni Paolo II sul balcone di San Pietro e disse all'Angelus*:* «Già troppo sangue polacco si è sparso per mani di polacchi nel corso di questo secolo. Basta con il sangue, con il metro del dialogo tutti i problemi possono essere affrontati e risolti». L'insurrezione che già era cominciata con scontri sanguinosi e violenti a Wadowice nelle miniere di carbone e in altre parti del Paese si fermò e tutti capirono che non ci sarebbe stata la temuta esecuzione degli ostaggi prelevati, che non sarebbe stato fucilato Walesa, che il Papa garantiva che non ci sarebbe stata effusione di sangue e che, d'altro canto, il dialogo avrebbe potuto cominciare. Per otto anni ci fu un dialogo difficile senza collusione con il potere, ma anche senza ricorso alla violenza e senza spargimento di sangue, se non da parte della polizia politica con l'assassinio di diverse persone, di cui il più noto è padre Jerzy Popieluszko. Siamo alle radici della ripresa della nostra libertà; l'Europa non si sarebbe costituita, l'allargamento non ci sarebbe stato, il quadro complessivo della difesa della pace nel mondo non sarebbe quello che è oggi, senza quella grande testimonianza. Voglio ricordarlo oggi in questo Parlamento e rivendicare il ruolo di quanti in Italia allora parteciparono appassionatamente a quella vicenda. Avrebbe potuto esserci una Bosnia-Erzegovina moltiplicata per 10, 20, 100 dal Baltico fino all'Adriatico; ci fu la capacità di contenerla, prima di tutto per quella grande testimonianza. Vorrei ricordare colui che allora fu il grande profeta di questa testimonianza: Giovanni Paolo II. In otto anni il più grande potere militare del mondo, il più grande apparato di oppressione poliziesca del mondo cadde non davanti ad una forza fisica fisica paragonabile, ma davanti ad una testimonianza intellettuale e morale. Credo che questo ancora debba essere oggi di insegnamento per ciascuno di noi. aver ricordato questo fatto rilevante per la storia dell'Europa. Come ha avuto la gentilezza di evidenziare, ricordo bene quella vicenda e credo di poter dire - oltre che sottolineare il mio apprezzamento per il suo intervento - che quando un popolo lotta per la propria libertà è un bene per tutta l'umanità e l'Aula non può che associarsi a questo ricordo. *(Applausi).*

*(AN)*. Signor Presidente, all'esame della 1a Commissione del Senato vi è l'Atto Governo n. 46, che è un decreto legislativo di recepimento di una direttiva dell'Unione Europea. Il termine per l'espressione del parere su questo decreto legislativo è stato fissato per il 21 dicembre, ma non è stata ancora calendarizzata la discussione del parere medesimo, benché sia all'ordine del giorno. Questo decreto legislativo, che riguarda una direttiva di 41 articoli, merita approfondimento e riflessione perché, oltre a realizzare una impropria parificazione tra tra convivenze e unioni matrimoniali, travolge e modifica nei fatti una serie di disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione e anche di norme antiterrorismo, che il Parlamento ha approvato con larghissima maggioranza poco più di un anno fa. Se non è stato ancora calendarizzato, o si presuppone una discussione molto veloce o addirittura - come in qualche caso purtroppo è avvenuto - si presuppone l'assenza di discussione, il che sarebbe veramente molto grave. È assurdo che vi sia un tale sovvertimento di norme importanti che reggono la nostra vita quotidiana senza un confronto ampio, e vorrei dire senza un confronto. La prego di sollecitare il Presidente della 1a Commissione alla più rapida calendarizzazione e alla fissazione di tempi che consentano tutti gli approfondimenti necessari per evitare che per via amministrativa o per via di recepimento di direttive comunitarie si eviti per l'ennesima volta il confronto democratico in questo Parlamento.

intervengo molto brevemente per associarmi alla richiesta del senatore Mantovano. Credo che l'incidenza che la direttiva in questione avrà su temi che saranno all'attenzione di questo Parlamento nei prossimi mesi impone la massima attenzione. Occorre non far passare questo parere nel silenzio, accreditando di fatto un meccanismo di silenzio-assenso che verrebbe a ledere le prerogative del Parlamento.

onorevoli colleghi, il dibattito sul bilancio che abbiamo svolto nella giornata di ieri è stato ovviamente intrecciato - inevitabilmente, come è prassi - a quello sulla manovra finanziaria.

tra DPEF, bilancio e finanziaria: credo che questo sia il punto vero. Dobbiamo avere la forza di affermare che il dibattito, come si è svolto, ha confermato che il bilancio di previsione per il 2007, come modificato dalla manovra correttiva proposta dal Governo, corrisponde pienamente agli obiettivi programmatici contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella relativa Nota di aggiornamento.

che io definisco strutturale e robusta perché il tema a cui ci richiamiamo è quest'idea di una manovra che coniughi in maniera contestuale, senza politica dei due tempi, rigore, equità e sviluppo; una manovra che volesse avere questa caratteristica non poteva basarsi solo su entrate fiscali, per altro non strutturali, ma doveva avere, una sua capacità di incidere sulla spesa e sugli investimenti produttivi: questo mi sembra l'aspetto importante. In terzo luogo, credo sia stato molto importante ed innovativo il dibattito sugli strumenti nuovi per il monitoraggio del Parlamento; è un dibattito cui ha dato un grande contributo il presidente Morando, ma che è riecheggiato anche in una serie di interventi. La mia proposta è che è necessario intervenire sul disegno istituzionale delle strutture che forniscono il supporto tecnico alle decisioni di politica fiscale; è necessario quindi avere uno strumento per il Parlamento tale da permettere, in corso di esercizio, attraverso un sistema di monitoraggio efficiente ed affidabile, un aggiornamento quasi in termini reali sia dell'andamento delle entrate, sia delle previsioni. Credo che sia giusto, come ha fatto il presidente Marini, intervenendo dopo il presidente Morando, chiarire che questa proposta parta dal Senato, anche se dovrà avere la capacità di coinvolgere anche l'altro ramo del Parlamento. Mi sembra che una struttura di monitoraggio sulle entrate e sull'andamento delle entrate fiscali

soffermarmi su alcune questioni. Mi sembra che tutti abbiano notato il tentativo, certo ancora insufficiente, di una trasparenza del bilancio che aiuti la comunicazione (io sono molto sensibile al tema della comunicazione). Da un lato, è evidente che dobbiamo auspicare di una sempre maggiore separazione fra indirizzo e controllo della spesa, che è il ruolo del Parlamento, e gestione della stessa. Il senatore Ferrara, anche qui, è intervenuto in maniera acuta su tale questione, ponendo il problema se sia opportuno o meno, in qualche modo, non tener conto del fatto che, all'interno di ciascun titolo di bilancio, sono rese possibili compensazioni di cassa da parte dei singoli Ministeri; con con un emendamento che come relatore ho apportato al disegno di bilancio, e che sarà al vostro esame fra qualche minuto, ho chiesto comunque di poterne informare le Commissioni parlamentari. Credo che sia una cosa giusta: non voglio fare polemiche, ma non avrebbe senso che il Parlamento debba essere implicato anche in piccole variazioni all'interno degli stessi capitoli. Anzi, il problema è esattamente l'opposto: di accentuare sempre di più una semplificazione che renda leggibile il bilancio sia per il Parlamento che per il Paese. Ecco perché ho accennato alla tematica del bilancio sociale, alla tematica del bilancio partecipativo. Da questo punto di vista, accanto al tema che ho posto del binomio flessibilità-riduzione della spesa (perché è stata, a me sembra, questa la tendenza degli ultimi anni: più si riduceva la spesa per una serie di Ministeri e di organi dello Stato, più si garantiva una qualche flessibilità per affrontare i problemi), bisogna porre un altro tema, e cioè quello della chiarezza delle priorità politiche: spetta al Parlamento dare chiarezza, spetta alle strutture attuarle, tenendo conto scrupolosamente delle priorità che, attraverso il bilancio e la legge finanziaria, il Parlamento definisce e potendo verificare in corso d'opera la coerenza fra

è in linea con le tre manovre di cui stiamo discutendo e di cui abbiamo discusso: il DPEF, la finanziaria, il bilancio stesso. Il tema della contestualità fra risanamento, equità e sviluppo è fondamentale. Credo che manterremo tranquillamente l'impegno in sede europea ad un rapporto fra indebitamento e PIL sotto il 3 per cento, andando probabilmente anche sotto il 2,8 per cento stimato all'inizio della manovra,

dobbiamo considerare che questo è il dato base dal quale è partita l'elaborazione sia della finanziaria che della legge di bilancio.

dovrebbe leggere qualunque documento di carattere comunitario o internazionale, qualunque previsione di agenzia o qualunque voce si sia levata su tale argomento per verificare che nessuno condivide tale timore. Oggi il maggior giornale economico d'Italia titola con la frase, limitata al settore industriale: «L'industria ritrova lo *sprint*». Noncredo che vi sia motivo per esultare e per dire che il nostro Paese abbia imboccato chissà mai quale strada, però è importante non aggiungere noi un effetto depressivo, spiegando che in realtà di fronte a un Paese che si sta riprendendo, e non necessariamente per volontà dall'attuale Governo ma anche per fatti obiettivi e per ragioni di carattere internazionale, non vi è alcuna ragione perché la classe dirigente politica dia al Paese un messaggio di tipo depressivo, che peraltro non è giustificato dai documenti di politica economica

Dicono anche, gli stessi giornali, la televisione, e si dice nei Palazzi e per strada, che il Governo sta ancora elaborando il testo del maxiemendamento. A questo punto, si tratterebbe di un ulteriore affronto al Parlamento che la prego di accertare perché con grande enfasi, e non con un Consiglio volante, è stata posta la fiducia su qualcosa che ancora non c'è.

In questa fase della discussione potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di emendamenti, per illustrarli, e quindi il relatore e il rappresentante del Governo per esprimere il rispettivo parere. Naturalmente sono ammesse le dichiarazioni di voto. Preciso che, con l'approvazione dei singoli articoli, si intendono approvati anche le Tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi del disegno di legge n. 1184, con le relative Note di variazioni.

Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole all'articolo 1, vorrei cogliere l'occasione per alcune riflessioni.

Sappiamo anche che c'è un affievolimento dell'importanza che questo strumento riveste ai fini di una programmazione e determinazione delle politiche di correzione dei saldi e di intervento sui fattori economici oggi affidati alla legge finanziaria.

del bilancio dello Stato finalizzata ad una rivalutazione dello stesso quale strumento autonomo di decisione politica nell'ambito della manovra politica

della politica economica dal versante delle entrate per il prossimo anno nonché di affrontare la questione

hanno portato ad un inasprimento permanente del prelievo fiscale nel 2006 per circa 3 miliardi.

a misure di carattere transitorio. Una particolare importanza ha avuto la riapertura dei termini per il versamento

l'aumento dell'imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni postali, l'imposta sulla riserva matematica delle assicurazioni. Tutto questo ha consentito

è dovuto in gran parte all'aumento dell'IRPEF, trainata dalla dinamica delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, ed è stato accentuato da quella progressività che le riforme fiscali della precedente legislatura hanno avuto sulla struttura di questa imposta. Questa progressività, infatti, è avvenuta in quanto non si è mai operato per la restituzione del drenaggio fiscale.

con quella che è stata una crescita molto contenuta per gli autonomi; nonostante la revisione degli studi di settore,

che le riforme varate dal centro‑destra hanno inciso duramente sul reddito dei lavoratori dipendenti. Aggiungo che è cresciuta fortemente anche l'IRES, circa del 20 per cento. Ma questo com'è avvenuto? È avvenuto perché, nella legge finanziaria per il 2006,

aspetti qualitativi. Quando sento i senatori dell'opposizione menare vanto di quello che è avvenuto nella passata legislatura, vorrei farli riflettere su come questa operazione

Aggiungo che il gettito dell'IVA, che invece è stato contenuto nei primi sei mesi dell'anno, sta crescendo moltissimo in questa seconda parte del 2006, per effetto delle iniziative, già prese dal Governo, che riguardano il controllo delle compensazioni ed un'azione decisa contro la frode fiscale dovuta all'«IVA carosello». carosello». Maggiore gettito, dunque, che nella seconda parte del 2006 ha altre caratteristiche, utilizza metodi di persuasione e di dissuasione ed introduce degli elementi di forte cambiamento. Cosa possiamo dire sulla politica fiscale fatta nella precedente legislatura? Parafrasando un detto celebre, possiamo dire che, nella passata legislatura (i dati confermano quello che è avvenuto), mai tanti hanno dato tanto per pochi. Ecco perché, nell'impostazione della finanziaria e della manovra della politica delle entrate, abbiamo questo segnale di cambiamento,

si esprimono con un'operazione di redistribuzione per quanto riguarda le aliquote dell'IRPEF, a sostegno delle famiglie e dei redditi medio bassi, e che si riferiscono ad un sostegno forte della ripresa dell'attività produttiva, riducendo la base imponibile legata al calcolo del lavoro dipendente per il sistema delle imprese, e ad un'azione forte contro l'evasione, l'elusione e

Signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo 1 per un semplice motivo che attiene anche alla funzione del bilancio. Uno dei principi del bilancio è quello della veridicità. L'articolo 1 non corrisponde più, allo stato attuale, a quello che ha affermato l'altro ieri il Vice ministro delle finanze; e dico «delle finanze» perché è rimasto un Ministero delle finanze, e poi vi è un Ministero del tesoro che è stato completamente assente nella discussione della finanziaria, sia alla Camera sia al Senato. Dunque, il Ministero delle finanze ha agito con reticenze, presentazioni, modifiche, errori marchiani, tabelle che non erano paragonabili un anno con l'altro, insomma con un metodo un po' oscuro, e dunque una certa reticenza, in Parlamento, c'è stata. Tuttavia il Vice ministro delle finanze, l'altro giorno, ha portato in Parlamento una tabella nella quale si dimostra come vi siano state delle cospicue entrate nel 2006, superiori, rispetto a quelle del 2005, non in misura banale ma nell'ordine di 34 miliardi di euro, quasi 70.000 dei vecchi miliardi di lire. ragionevolezza vorrebbe che, se non altro per chiarire l'entità di queste entrate, il Governo presentasse una Nota di variazioni per iscrivere in bilancio tale crescita, cosa che non è stata fatta.

di dire più avanti. Questa operazione-verità non è stata fatta per la semplice ragione che se noi facciamo emergere esclusivamente le entrate, poi siamo necessitati a confrontarci con tale emersione e a valutare il livello di spesa che poi si propone con la finanziaria; se invece portiamo tutto nel medesimo calderone, poi creiamo un regime di nebbia e di confusione dal quale non è lecito e non è chiaro capire come la finanziaria muova i flussi sia in entrata sia in uscita. ha detto poco fa il vice ministro Pinza, queste maggiori entrate non comportano necessità di diminuire la manovra perché la manovra non è recessiva. Questo non è vero, signor Vice ministro, basta leggere la relazione previsionale e programmatica che avete scritto voi, basta leggere la Nota integrativa del Documento di programmazione che avete scritto voi, per vedere come il 2007 subirà gli effetti recessivi di questa manovra e il tasso di sviluppo dello stesso anno sarà inferiore rispetto a quello di sviluppo tendenziale, al netto della manovra, ognuno è figlio dei propri mali e questo sarà il primo effetto. Il secondo effetto, signor Presidente, è che con questo livello di confusione delle entrate si può mascherare, ed è quello che ha fatto il Governo, la manovra di spesa facile che è stata fatta con questa finanziaria perché

trasmesso al Parlamento contiene elemosine per circa 1 miliardo e 600 milioni di euro; la Camera ha aggiunto i famosi accordi politici per circa 700 milioni di euro e il motivo per cui ritardano i nostri lavori (non so se il maxiemendamento sarà presentato alle 12, alle 13, alle 17 o alle 18, e non importa sotto questo profilo), il motivo per cui abbiamo ritardato in Commissione e la Commissione non è riuscita a chiudere i lavori, e il motivo per cui il Senato sta aspettando i comodi dei signori della maggioranza, è che essi si stanno squartando su circa un miliardo di spese aggiuntive ulteriori che non va certo a risanamento del Paese, ma serve a coprire gli appetiti di questo o quel Gruppo politico marginale che minaccia, senza ovviamente averne la forza (ma qui si evidenzia la forza del Governo che, minacciato, com'è stato molto spesso, con pistole ad acqua, si è sempre arreso in questa vicenda politico finanziaria), di non votare la finanziaria se non sarà accontentato. Il risultato è che i contribuenti italiani dovranno pagare circa un miliardo di euro in più per le domande che voi signori della maggioranza volete inserire nel testo attraverso emendamenti la cui portata non è sicuramente di storico rilievo in questa finanziaria. nuove entrate non vengono evidenziate con chiarezza è esclusivamente quello di confondere le acque e consentirvi di portare avanti questa politica clientelare e di basso governo

di questa finanziaria che non determina variazioni sulla linea di povertà delle famiglie. Questo è il dato: non vengono tenuti in considerazione né i pensionati né gli incapienti. Questi sono risultati scientifici che devono essere Per queste ragioni, Presidente, chiediamo la pubblicazione di questa tabella ed al tempo stesso votiamo contro questo articolo.

3 per intervenire anche su alcuni temi posti alla nostra attenzione dai colleghi, in particolare, da ultimo, dal senatore Vegas. Il nostro bilancio registra, in effetti, una congiuntura positiva della nostra economia: una forte riduzione del saldo netto da finanziare, un marcato miglioramento del risparmio pubblico, un conseguente incremento dell'avanzo primario. È una fotografia a nostro parere nitida e confortante, ma, essendo appunto una fotografia, non può per definizione cogliere tutti i cambiamenti intercorsi dopo lo scatto. Da una decina di giorni l'opposizione denuncia una volontà governativa volta ad occultare la realtà. In particolare, sarebbe in corso un'operazione mistificatoria atta appunto ciò che è vero sull'ottimo andamento delle entrate fiscali nell'anno 2006. Quella descritta dalle opposizioni si configurerebbe quindi come un'operazione sofisticata, lungimirante, basata su una capacità di analisi e previsione di altissimo livello, il tutto poi al servizio di una volontà politica volta ad accumulare di nascosto risorse aggiuntive da utilizzare successivamente. Questa ipotesi ci sembra francamente esagerata e infondata. Più modestamente riteniamo che il Governo è stato guidato da un criterio di prudenza forse eccessivo, ma, visto anche ciò che è successo in questi mesi (sentenza europea sull'IVA relativa alle auto) e considerato che il forte aumento delle entrate fiscali va parametrato non tanto sulle entrate del 2005 ma sulle previsioni della precedente finanziaria, e quindi che il margine il margine è assai minore rispetto a quello che oggi viene descritto, e considerato anche ciò che leggiamo questa mattina sui giornali circa successivo rallentamento di alcune ipotesi di entrata, credo che questa prudenza da parte del Governo vada considerata positivamente. Per tale ragione voteremo favorevolmente a questo articolo.

Il bilancio che esaminiamo prevede, nello stato di previsione, spese correnti per competenza, per autorizzazioni di cassa, in conto capitale e per dimensioni di interventi appunto sulla cassa. Il rimborso delle passività finanziaria ammonta a 189 miliardi di euro e le risorse complessive sono pari a 450,7 miliardi di euro di competenza e a 462 miliardi di euro per le autorizzazioni, con una significativa riduzione rispetto all'assestato 2006 (circa 10 miliardi), a dimostrazione del sforzo di contenimento della spessa corrente complessiva. Nel quadro di questo generale apprezzamento per le diverse autorizzazioni di spesa prefigurate nei vari commi di cui si compone l'articolo mi limiterò ad alcuni peculiari elementi di sottolineatura per le parti che hanno formato oggetto delle valutazioni del nostro Gruppo e della maggioranza in Commissione finanze. fare riferimento al centro di responsabilità relativo alle politiche fiscali, che registra rispetto al dato assestato 2006 un incremento di competenza significativo, a dimostrazione, con questo cinque per cento di incremento della spesa corrente, dello sforzo che la manovra di bilancio 2007 dispiega sia per rafforzare il funzionamento delle diverse strutture preposte all'attuazione di più efficaci politiche fiscali sia per dare impulso a più ampie azioni perequative e redistributive, oltre che di incentivazione tramite diverse modalità di agevolazione fiscale e contributiva alle imprese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Anche la Guardia di finanza, rispetto al dato assestato del 2006, registra un incremento di spesa in termini di competenza, passando dai 3.416 milioni delle previsioni assestate a 3.521 milioni delle previsioni del 2007. Con l'occasione formulo l'auspicio che nel maxiemendamento, che il Governo si accinge ad adottare, siano racchiuse anche altre ulteriori provvidenze, in generale per tutti gli impegni relativi al cosiddetto pacchetto sicurezza. impegni - lo sottolineo - che hanno costituito oggetto di una positiva concertazione con la stragrande maggioranza dei sindacati rappresentativi (circa il 90 per cento degli operatori di polizia, oltre quelli della Difesa e di altri quattro Ministeri). Qui, in particolare, limitandomi al ragionamento sulla Guardia di finanza, vorrei evidenziare la delicatezza e l'importanza di attrezzare con adeguate dotazioni finanziarie l'operatività della stessa che proprio in aderenza agli obiettivi di lotta all'evasione ed elusione fiscale, convintamente perseguiti dal Governo e dalla maggioranza, sarà chiamata ed è chiamata ad ampliare la propria attività di istituto su fronti decisivi e quanto mai sofisticati come sono, ad esempio, quelli della tutela degli interessi erariali nel settore delle frodi e della lotta alla contraffazione. In questo quadro va giudicato di particolare rilevanza il potenziamento del sistema antifrode, di cui alla legge n. 166 del 2005, imperniato sull'attività dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento che esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi riguardo ai pagamenti dilazionati o differiti effettuati attraverso la rete *internet* ovvero relativi al settore assicurativo. In questo campo, si registra negli ultimi tempi un vero *boom* di truffe ai consumatori e di frodi verso il fisco e occorre, per potenziare le capacità di contrasto al fenomeno, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa agire con più poteri di riorganizzazione e rafforzamento degli uffici preposti. In conclusione, vorrei fare due brevi considerazioni generali, riprendendo spunti emersi da una discussione in Commissione che non hanno purtroppo potuto trovare sviluppo nell'adozione compiuta di un parere formale, ma sono tuttavia ben meritevoli di essere rappresentati come elementi di giudizio rafforzativo del nostro voto positivo. Mi riferisco al tema della valorizzazione del patrimonio pubblico, per com'è affrontato nella manovra di bilancio e poi in quello che al momento è l'articolo 18, comma 13, della finanziaria, laddove si prevede l'attivazione di programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali presenti in un determinato contesto territoriale. In particolare, sottolineo la facoltà che viene riconosciuta all'Agenzia del demanio di individuare una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico e organicamente formulato con il concorso dei soggetti istituzionali del territorio interessato. Con le norme in questione si interviene poi per razionalizzare e coordinare disposizioni non sempre coerenti intervenute negli ultimi anni in materia di dismissione degli immobili in uso all'amministrazione della Difesa, rimuovendo gli ostacoli che, in alcuni casi, hanno impedito la piena attuazione del processo di dismissione. La finalità complessiva della nuova impostazione è invece proprio quella di ricondurre in un'unica procedura la dismissione degli immobili in uso all'Amministrazione della difesa, dando con ciò finalmente prospettiva di concretizzazione (che mi piace ricordare anche per aver avuto occasione di trattare e risolvere con lui quella che credo sia rimasta una delle poche transazioni felicemente concluse),

Da ultimo, vorrei ribadire, ricollegandomi alle importanti considerazioni svolte ieri in Aula dal senatore Morando, che è stato anche un convincimento unanime, condiviso in Commissione e autorevolmente sottolineato nel corso della discussione proprio dal presidente Carlo Azeglio Ciampi,

consentendo inoltre ai Gruppi politici e ai singoli parlamentari di concentrare la loro attenzione sulle linee di fondo e sulle scelte fondamentali di politica economica, anche per rendere più visibile e giudicabile l'alternatività di proposte tra maggioranza e opposizione. In questa prospettiva potrebbe essere opportuno e utile prevedere una relazione governativa, in sede di presentazione alle Camere del progetto di bilancio e della legge finanziaria, sullo stato di attuazione della stessa legge per l'anno in corso, ferma restando la disciplina del rendiconto e dell'assestamento di bilancio e delle relazioni al Parlamento sugli andamenti della finanza statale. Questo, voglio dirlo, è un elemento di innovazione che si può fare a legislazione vigente - noi ci auguriamo anche altre modificazioni - ed è augurabile che possa essere proposto già dal prossimo anno da parte del Governo, anche per dare conto - mi auguro - degli effetti positivi che, dalle scelte del bilancio e della finanziaria 2007, contiamo deriveranno all'economia e alla società italiana. Signor Presidente, dichiaro preliminarmente la nostra volontà contraria all'approvazione dell'articolo 3. 3. Vorrei poi richiamare l'attenzione dell'Aula e di tutti i colleghi, perché probabilmente le prime ore del mattino non ci lasciano intendere cosa stiamo realizzando in quest'Aula. Stiamo discutendo per approvare il bilancio dello Stato; il bilancio dello Stato è una legge formale, dovrebbe contenere soltanto numeri, ha invece all'interno disposizioni e di questo ci siamo dilettati a parlare noi dell'accademia, della Commissione bilancio. su un articolo che ha un contenuto squisitamente e specificatamente formale, abbiamo l'opposizione che ha fatto mezz'ora di intervento, il senatore Barbolini ha superato se stesso, ha fatto tutte le citazioni possibili e immaginabili, citato il grande presidente Andreatta che sull'approvazione dell'articolo 3, in questo momento, non c'entra nulla, perché anche lui sarebbe scandalizzato, se fosse in quest'Aula, di come stiamo evolvendo la discussione sul bilancio dello Stato, legge formale. Allora, cortesemente, signori della maggioranza, finitela di fare opposizione a voi stessi; se il maxiemendamento non è pronto, sospendiamo questa seduta, potremmo restituire i Ministri al loro lavoro, anche se di questo non siamo contenti perché, quando lavorano, lavorano male per il Paese. Potremmo restituire il presidente Marino e il ministro Turco ad un lavoro che li sta vedendo fitti fitti parlare, perché dell'Aula non gliene importa niente. Un attimo di serietà allora! Sospendiamo la seduta, così come abbiamo fatto ieri, perché non siete pronti! Questa è una comica e avete votato in Consiglio dei ministri una fiducia prescindendo - come diceva Totò - perché siete dei comici e non delle persone serie!

evitare questo brusìo perché è veramente difficile parlare. RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, siamo in sede di votazione e credo che sia difficile sospendere la seduta, eventualmente la Presidenza deciderà dopo, quando avremo finito di votare. Personalmente, ritengo che dobbiamo continuare i nostri lavori, come avremmo dovuto continuarli ieri. Utilizzo questa occasione annunciando il voto favorevole su un articolo formale - come ha detto il senatore Ferrara per esplicitare la nostra posizione su una questione formale, posta dall'opposizione, circa la necessità di procedere alla Nota di variazioni del bilancio per recepire le maggiori entrate che si sono verificate in questi ultimi mesi. mesi. L'opposizione ha posto l'attenzione su questo problema dicendo che è merito della politica economica e fiscale del Governo precedente, il fatto che in questi mesi si sia verificato un aumento consistente del gettito. Ovviamente, non posso negare questa che è una verità; a legislazione vigente, quindi a fronte delle leggi varate dal Governo precedente, c'è stato e c'è un aumento della pressione fiscale. Tuttavia, credo che l'opposizione debba convenire con noi

Se si vuole definire a chi spetta il merito, quantomeno dovremmo attribuirne una parte al vecchio Governo e una parte alle politiche adottate dall'attuale Governo. Circa la consistenza delle maggiori entrate e la necessità, affermata dall'opposizione, di procedere ad una Nota di variazioni al bilancio,

procedere alla Nota di variazioni del bilancio credo rappresenti una decisione affrettata. Infine, signor Presidente, voglio ricordare che in queste ultime settimane sono stati accertati ulteriori

Signor Presidente, l'articolo 7 e la tabella 7 del bilancio per il 2007 descrivono l'intervento sull'istruzione, *(Ulivo)*. L'articolo 7 descrive l'intervento sull'istruzione, il quale opera già scelte strategiche. Ricordo che esaminiamo, in Aula, questa parte del bilancio dopo che ne abbiamo parlato in un ampio ed approfondito confronto, anche con l'opposizione, nella 7a Commissione, come come è avvenuto anche nella Commissione bilancio. Parliamo del Ministero della pubblica istruzione dopo la sua nuova riorganizzazione, a seguito dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 181 del 2006. A tale Ministero sono attribuiti 22 centri di responsabilità amministrativa così suddivisi: al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, sul quale, voglio ricordare, sono operati tagli per il contenimento dei costi della politica; al Dipartimento per la programmazione ministeriale e il bilancio, al Dipartimento per l'istruzione ed agli uffici scolastici regionali. Voglio notare che l'incidenza percentuale sul totale del bilancio dello Stato è pari circa al 9,2 Vi è un incremento, nel bilancio per il 2007, di 967,2 milioni di euro rispetto all'assestamento per il 2006 ed un aumento del 2,3 per cento, mentre nel 2006 si era verificata una riduzione, rispetto al 2005, dell'1,6 Dunque, questo è il primo segno del cambio di Governo, è il primo bilancio del Governo dell'Unione e la prima assunzione di responsabilità sul presente del Paese per il suo futuro sul terreno, delicatissimo e strategico, dell'istruzione. Rilevo che l'incremento rispetto al bilancio 2006 è pari al 5,7 mentre si registrava nel 2006 una diminuzione, rispetto all'anno precedente, dell'1,6 per cento. Si registra inoltre, nel bilancio 2007, un decremento dei residui passivi rispetto all'esercizio 2005; è il primo segnale, dunque, del miglioramento del quadro finanziario per l'istruzione rispetto agli anni precedenti. Il secondo segnale è una scelta storica che apre una nuova fase nella gestione finanziaria dell'istruzione: l'articolo 7 del disegno di legge di bilancio precisa che il Ministero dell'economia, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire i fondi, nell'ambito delle unità previsionali di base, secondo due canali precisi e ben distinti: il primo, i fondi da ripartire per oneri di personale; il secondo, i fondi da ripartire per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, cioè per l'operatività scolastica. Con quest'ultimo fondo, la finanziaria approvata alla Camera dispone, al comma 261, la diretta allocazione delle risorse per due miliardi e 800 milioni alle istituzioni scolastiche secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro senza vincoli di capitoli e, quindi, con la totale responsabilizzazione di spesa delle istituzioni scolastiche e l'avvio del monitoraggio delle spese effettuate dalle scuole. È la scelta storica di finanziare l'autonomia delle istituzioni scolastiche già definita dalla nostra Costituzione. Infatti, è necessario sapere, e si sa,

delle sezioni delle scuole dell'infanzia dai due ai tre anni, l'innalzamento dell'obbligo a sedici anni, il piano dell'educazione per gli adulti, rivolto in particolare agli immigrati, la formazione tecnica superiore, le attrezzature tecnologiche, l'edilizia scolastica, la messa in sicurezza degli edifici, la scuola aperta al territorio per combattere violenza e dispersione, il finanziamento delle scuole paritarie, in particolare Su questo articolo e su questa tabella si giocano il senso dell'autonomia con l'obiettivo strategico della qualità e della verifica dei risultati. Da questo punto di vista, c'è l'investimento nuovo

se si indicano obiettivi di risultati, se si applica una collaborazione forte tra Stato, Regioni, enti locali, istituzioni scolastiche e se si ha il coraggio di una vera valutazione dei risultati, di un controllo e di un monitoraggio delle spese. Il bilancio del Ministero della pubblica istruzione mostra che questo è solo il primo passo perché occorrono certamente più risorse ma occorre, innanzitutto, la consapevolezza politica del cambio di passo. Questa consapevolezza il Governo l'ha espressa. Occorre procedere su questa strada perché scegliere l'autonomia significa, appunto, valutare i risultati; incrementare su questa base le risorse per fare crescere la qualità dell'istruzione e, attraverso l'istruzione, rimettere in moto il Paese.

che occorre una programmazione politica sul governo del personale della scuola, sugli esodi, sulle assunzioni, sull'esaurimento delle graduatorie del precariato, su un nuovo reclutamento per l'istruzione

che seleziona gli obiettivi, cancella gli sprechi, investe davvero sul futuro, cambiando lo stato delle cose con due strumenti:

chiedendo semplicemente la fedeltà alla missione pubblica della scuola nazionale. È il ruolo della politica per il futuro dell'Italia che già intravediamo tra i conti al nostro esame.

che, offendendo me e in me il Senato, non ha risposto alle mie interrogazioni, ma mi ha fatto rispondere attraverso il vero Ministro dell'interno, che è il Capo della Polizia, attraverso un oscuro funzionario suo servitorello, capo di un sindacato inesistente di cui il Capo della Polizia si è servito per cercare di fiaccare i sindacati veri. Una di queste interrogazioni era particolarmente delicata perché con essa chiedevo al Ministro dell'interno se il Capo della Polizia - che sa tutto sapesse dell'azione, per la quale l'ho denunziato alla procura di Brescia e per cui è in corso l'inchiesta di quella stessa procura, di spionaggio sulle persone, sulle sedi e sulle comunicazioni telefoniche del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare e se, sapendolo, ne abbia informato il Ministro dell'interno dell'epoca. Se ha detto di non sapere, come capita sempre, il prefetto De Gennaro è un grande mentitore e, se sapeva e non ha informato il Ministro dell'interno, è un infedele. Voto contro finché a quel posto ci sarà un losco figuro come il prefetto De Gennaro, servitorello del *Federal Bureau of Investigation*, al quale ha fatto sporchi servizi, perseguitando nel processo di Palermo uno degli uomini più importanti del partito di cui io mi sono onorato di appartenere: la Democrazia Cristiana.

di grande significato per gli argomenti che ha introdotto in Aula. Credo che di fronte denunce così gravi il Senato non possa

delle quali ovviamente - lo dico in maniera del tutto tecnica - si assume la responsabilità perché non è dato sapere se ...

segreto che non è in grado di agire e può essere intercettato come e quando fare l'autorità giudiziaria e di cui non si fida più nessun servizio segreto del mondo occidentale, con la conseguenza che non riceve più notizie essendo ormai assolutamente trasparente. Su questo tema il Ministro della giustizia *pro tempore* - non è questione di nomi, ma di funzione - ha la possibilità di addivenire alla richiesta di arresto avanzata per alcuni personaggi stranieri. In passato io non lo feci avvalendomi delle prerogative di legge e considerando che, per la sicurezza dello Stato, non si poteva arrivare a questa richiesta di arresto. Sono stato criminalizzato in sede nazionale ed internazionale, ma vedo con piacere che oggi il ministro Mastella segue esattamente le mie orme.

Senatore Matteoli, le di ascoltare in un'Aula parlamentare una denuncia così forte e netta da parte di un autorevole membro di questa Assemblea. Credo che il Senato non possa fare a meno di registrare ciò che ha detto il senatore Cossiga e di chiedere al Ministro dell'interno di venire in Aula a riferire. a riferire. Assistiamo in questi giorni ad un balletto di arresti e liberazioni che lascia perplessi tutti i cittadini:

C'è una denuncia molto forte, per cui auspico che il Governo voglia venire a riferire e che il Ministro dell'interno venga in quest'Aula a confutare

di un autorevolissimo ed anziano senatore, che, appunto per quest'ultima qualità, se non dovesse essere ascoltato, sarebbe anche offeso. Questo è il Senato della Repubblica; Cossiga ha denunciato più volte una vicenda di tale gravità. Siamo anche in ritardo rispetto all'esigenza di conoscere, da parte della Camera alta, la verità; che il ministro Amato, raccolta la documentazione, venga finalmente a riferire in Aula. Vorrei aggiungere un'altra considerazione. Sto preparando un'interpellanza urgente al Ministro della della giustizia - che è presente in Aula - per conoscere se è prevista, dalla legislazione italiana, la possibilità di usare tortura verso i detenuti. Ci sono molte forme di tortura; in questo Paese, più volte, una di queste è stata utilizzata. Signor Ministro, vorrei sapere - e lo metterò per iscritto - se in questo Paese è possibile far rispettare la legge anche da parte di alcuni magistrati.

la prima volta che ascoltiamo le parole del presidente Cossiga su un argomento così delicato; non è la prima volta che ascoltiamo, da parte di un ex Capo dello Stato, che rispettiamo, delle accuse non indifferenti, rese in quest'Aula. Noi non intendiamo - né abbiamo titolo per farlo - entrare nel merito della veridicità, della bontà della fondatezza di queste considerazioni. Vi è però un dato istituzionale: un'esigenza di ascolto, da un lato, e un'esigenza di non indifferenza al chiarimento su questi temi, dall'altro. Una non indifferenza all'obbligo del Governo a riferire e a rispondere alle accuse che il presidente Cossiga oggi ha ritenuto di dover ripetere in questo consesso, nel momento in cui esso è riunito nella sua totalità ad approvare il disegno di legge finanziaria; in una seduta, quindi, che già di per sé, per l'argomento che tratta, si presenta come seduta sicuramente autorevole, sentita e seguita dall'intero Paese. Abbiamo un dovere: noi, come opposizione, lo stiamo esercitando con serenità e pacatezza, attraverso gli interventi dei Capigruppo, nel chiedere al Governo di venirci a rassicurare, quanto meno, su come stanno le cose. Abbiamo assistito, in questi anni, ad una crescita della nostra *intelligence;* attraverso la nostra *intelligence* abbiamo ottenuto dei risultati non indifferenti nel contrasto al terrorismo, nel contrasto ai rapimenti di nostri italiani in territori iracheni ed altro. La nostra *intelligence*, in questi anni, ci ha abituato ad essere orgogliosi del suo lavoro, realizzato in tutta la mappa mondiale. Allo stesso tempo, all'interno del Paese si susseguono eventi e momenti che ci preoccupano: arresti, scarcerazioni, inchieste, controinchieste. Vi è una certa preoccupazione, che avvertiamo e che vorremmo scongiurare. Noi abbiamo, secondo me, come Italiani il diritto‑dovere di essere orgogliosi dei nostri servizi e il diritto-dovere di sapere cosa c'è di male, di strano, di ammalato - se c'è - all'interno dei nostri servizi e dei nostri apparati. Quindi, l'appello del presidente Cossiga, secondo noi, non può e non deve essere lasciato inascoltato, ma deve servire affinché il Ministro dell'interno venga

a nome del Gruppo al quale appartengo devo dire che anche noi riteniamo che sia arrivato il momento che il Governo e il Ministro dell'interno dicano una parola chiara su questa vicenda. Per la seconda volta in quest'Aula un'autorevole personalità della Repubblica italiana ha sollevato un problema che è innanzitutto istituzionale. Egli da tempo ha chiesto al Governo, con un'interrogazione, di rispondere rispetto ad un'ipotesi sulla quale, ovviamente, non entro nel merito, ma che comunque si configura come una dura denuncia nei confronti di chi ha oggi responsabilità rilevantissime nell'interesse dei cittadini, e cioè il Capo della Polizia. il Capo della Polizia. La risposta sarebbe dovuta a qualunque parlamentare, ma il senatore Cossiga, nella sua autorevolezza e nel suo convincimento, ha posto la richiesta più volte, ha preannunciato anche le sue dimissioni da senatore oggi vota su questo punto, a differenza dell'opinione che ha fin qui liberamente espressa contro il Governo sulla tabella del Ministero dell'interno. Ripeto: il Ministro dell'interno ha il dovere non di dare ragione al senatore Cossiga, ci mancherebbe altro, ma

Anche noi ci associamo alla richiesta, fatta dal senatore Matteoli in particolare, che vi sia una seduta esplicitamente dedicata alla risposta politica del Ministro dell'interno nella quale si possa anche capire per quale motivo, per la prima volta nella storia dell'FBI, è stato dato un riconoscimento al prefetto De Gennaro. Quindi, vorremmo che tutta la vicenda potesse essere oggetto di un dibattito parlamentare in Aula. Non credo che la bocciatura dell'articolo del bilancio che riguarda il Ministero dell'interno possa rimanere, per così dire, senza traccia, perché sarebbe una reazione eccessiva. Noi voteremo contro, come abbiamo votato contro complessivamente il bilancio per ragioni politiche,

Presidente, a nome del Gruppo Verdi- Comunisti Italiani vorrei appoggiare la richiesta avanzata. Credo che sia una questione che richieda grande senso di responsabilità per Aula e soprattutto per il Paese. Noi dobbiamo rassicurare il Paese, dobbiamo chiarire, dobbiamo impedire soprattutto che si alzino polveroni. Appoggiamo quindi la richiesta rivolta al Ministro dell'interno. il Parlamento ha il dovere di rassicurare il Paese attraverso le risposte che dovranno essere fornite al senatore Cossiga.

Penso che il senatore Cossiga abbia sollevato un problema delicatissimo che riguarda non un cittadino qualsiasi, ma un elemento fondamentale per l'andamento dello stato dell'ordine pubblico come il Capo della Polizia e credo sia giusto che il Ministro dell'interno venga a riferire in Parlamento sulle vicende che il senatore Cossiga ha denunciato nell'interrogazione e poi in due suoi interventi. Detto ciò, aggiungo che che starei attento ad una riflessione troppo semplificata sulle vicende che riguardano i servizi di *intelligence* nel nostro Paese.

Presidente, colleghi, il Gruppo Per le Autonomie non vuole entrare nel merito della questione, però sottolinea quanto già evidenziato dai colleghi. Mi sembra un atto dovuto, un atto di rispetto nei confronti del senatore Cossiga, Cossiga, oltre che un atto dovuto verso il Parlamento intero, che il Ministro dell'interno si faccia carico di una risposta chiara e veloce al Parlamento

che riguardano l'essenza della funzionalità di un qualcosa che, per essere un Servizio, per giunta segreto, ha il dovere-diritto di un'estraneità ad altri rapporti, ad altre situazioni, per una valutazione di interessi superiori che possono essere considerati prevalenti. Dice il senatore Cossiga: io voto contro. Io, invece, chiedo che sia accantonato l'articolo 8 e che il Ministro venga subito a riferire; dopodiché, potremo votare tale l'articolo con sicurezza: ci si salva poco l'anima votando contro, avendo sempre finora votato a favore! Questo è quanto dico io. È la mia opinione, non so se condivisa dal mio Gruppo. Ma proprio

il compito di stabilire se il dovere di appartenenza debba essere superato dai doveri della coscienza. Quando sento dire che il Capo della Polizia è un losco figuro, ho il diritto di sentire dal Ministro un sì o un no e prima di votare una tabella, ho il desiderio di ascoltare la parola del Ministro. Chiedo, pertanto, l'accantonamento della votazione dell'articolo 8, fino a quando il Ministro non avrà risposto in Aula.*(Applausi

Credo che il senatore Biondi abbia fatto una richiesta politica di rilevante importanza. Il dibattito suscitato dalla richiesta del senatore Baldini a seguito delle dichiarazioni del presidente Cossiga

non vi è la votazione dell'Aula, come accadrebbe alla Camera, ma è nella facoltà del Presidente di verificare se esistono le condizioni; probabilmente, si può anche, via informale, accertare se vi è una disponibilità del Ministro dell'interno e decidere quando, eventualmente, votare. Però, non sottovaluterei l'importanza della richiesta politica del senatore Biondi.

di una vastità di opinioni che mi sono apparse convergenti su quanto espresso dal senatore Cossiga, senza entrare nel merito, peraltro pur nella collegialità e nella responsabilità del Governo e per non dare l'idea di un Governo assente rispetto al dibattito,

ringrazio, Ministro. Mi pare che le considerazioni ed i chiarimenti del Governo siano, almeno per la Presidenza, sufficienti ad assicurare, rispetto all'andamento del dibattito e alle sollecitazioni

capitale aumenta dopo che negli anni scorsi si era registrato l'esatto contrario. Le politiche del passato Governo, com'è noto, avevano sospinto la spesa corrente verso un incremento vertiginoso: fino al 3 per Aumenta il fondo per le opere strategiche, aumentano i fondi per interventi vari (Venezia, Roma capitale, opere stradali, trasporto rapido di massa molti altri interventi sono poi previsti per il trasporto e per il trasporto pubblico locale), ma i dati che si evincono dalla tabella all'articolo 10 sono destinati ad accrescersi se, come tutti ci auguriamo, nel maxiemendamento del Governo saranno accolti gli emendamenti che lo stesso Governo ha presentato ed illustrato in Commissione bilancio durante l'esame della legge finanziaria. Da tali emendamenti e dall'intervento del Ministro dell'economia, sempre in Commissione, si evince in via definitiva il carattere propagandistico delle politiche infrastrutturali degli anni scorsi, che si sono arrestate alla rappresentazione grafica, per così dire, esternata in via televisiva nei modi e nei tempi che tutti noi ricordiamo. evidenziare una tabella che il Ministro ci ha presentato in Commissione, sintomatica delle affermazioni che ho appena fatto e che è utile che l'Aula esamini e tenga in debito conto. Mi riferisco a quella relativa alle risorse attribuite all'ANAS e alle Ferrovie. Il Ministro ci ha riepilogato alcuni dati significativi: le risorse attribuite ad ANAS nel 2004 erano pari a 2 miliardi e 593 milioni di euro; nel 2006 sono state di 1 miliardo e 440 milioni di euro: un dimezzamento delle risorse per investimenti infrastrutturali affidati ad ANAS. Siamo dovuti intervenire con 1 miliardo di euro con il decreto Bersani e con ulteriori 289 milioni di euro con la legge finanziaria al nostro esame, cosicché le risorse complessivamente attribuite quest'anno ad ANAS sono ritornate a crescere fino a 2 miliardi e 989 milioni di euro, una cifra superiore a quella del 2004. Ancor più significativo è il dato delle ferrovie: dai 5 miliardi e 779 milioni di euro del 2004 si è scesi vertiginosamente nel 2006 a 2 miliardi e 968 milioni. milioni. Anche qui il Governo è intervenuto con 1 miliardo e 800 milioni con il decreto Bersani e con ben 3 miliardi e 623 milioni con la legge finanziaria, riportando il dato delle risorse per Ferrovie a 6 miliardi e 748 milioni di euro, un dato di molto superiore a quello del 2004.

che certamente sarà incluso nel maxiemendamento per le ragioni che esporrò fra poco. Esso considera appunto la situazione che è venuta a determinarsi il finanziamento dell'alta velocità e dell'alta capacità. La legge finanziaria per il 2003 ha introdotto un meccanismo di finanziamento del sistema ad alta velocità da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, la TAV-RFI, basato su prestiti concessi allo stesso gestore da Infrastrutture S.p.A., che poi è stata fusa con la Cassa depositi e prestiti. Si tratta di un fondo che si è finanziato con il ricorso al mercato dei capitali. Il rimborso di questi prestiti avrebbe dovuto essere assicurato dai flussi di cassa generati nel periodo di sfruttamento economico dell'opera, ma così non è avvenuto perché l'infrastruttura non è completata e questi questi rientri non si sono verificati. Nel maggio del 2005, EUROSTAT ha riclassificato le passività di ISPA, che erano state tenute fuori

EUROSTAT. Con l'emendamento che ho sopra menzionato, pertanto, si è provveduto a questa riclassificazione per una cifra che ascende a 12 miliardi e 900 milioni di euro, dunque quasi 13 miliardi di euro che sono confluiti sull'ammontare del debito pubblico e che hanno inciso, unitamente al debito pregresso per IVA, per 17 miliardi sul disavanzo, facendo balzare il *deficit* del 2006 dal 3,6 per cento che era stato rilevato al 5,7 per cento, come rilevato in data di ieri con l'aggiornamento del programma di stabilità redatto dal Governo.

gli interventi che saranno esaminati e che sono stati già previsti sia nel testo licenziato dalla Camera sia negli emendamenti del Governo che riguardano la Pedemontana

E non sto qui a citare molte altre voci di investimenti, per esempio nella sanità, nell'edilizia universitaria, nella difesa. Insomma, si ricomincia con una politica infrastrutturale seria, basata non sulle chiacchiere, sui pedaggi ombra, sulla finanza creativa, ma su scelte concrete e denaro vero. Questa finanziaria, signor Presidente, anche per queste ragioni, è migliore di quanto si è fino a questo momento ritenuto. Anche per tale motivo, dichiaro il nostro voto favorevole all'articolo 10.

Presidente, l'interruzione degli interventi dei colleghi della maggioranza, poc'anzi, mi aveva fatto intuire, costruendo un processo deduttivo alla Sherlock Holmes, che era arrivato il testo del maxiemendamento. Poi, invece, hanno ripreso a parlare e a questo punto ho capito che c'era stato un «contrordine, compagni». Tuttavia, quello che non capisco è il motivo per cui una persona autorevole e componente della Commissione bilancio, come il senatore Legnini, si debba inventare un intervento di questo tipo che non ha nulla di scientifico. tipo che non ha nulla di scientifico. Stanno intervenendo sul bilancio perché probabilmente faremo una discussione molto più contenuta sulla finanziaria e allora qualcuno vuole intervenire adesso sul bilancio. Ma, in questo senso, mi aspetterei allora che parlassero della finanziaria, invece continuano a parlare del bilancio.

delle connotazioni di falsità e quindi, invece di parlare di cose false, se debbono perdere tempo, potrebbero anche parlare di sport, tanto il tempo glielo lasciamo perdere lo stesso, per evidenziare il modo con cui questa maggioranza sta facendo opposizione a se stessa. Il senatore Legnini dice il falso per tre motivi principalmente. Uno: è inutile che parla della TAV e degli aumenti dei fondi disponibili per l'ANAS, perché codesto Governo, rosso-verde, sulla TAV aizza gli amministratori locali, i sindaci e se stesso contro tutto e tutti; non ha nessuna intenzione di farla. Due: perché ciò che dice sull'EUROSTAT è completamente inventato, perché si legge assolutamente il contrario nei documenti che sono già da tempo tra gli atti parlamentari a nostra disposizione e in merito ai quali si è fatta lunga discussione in Commissione.

nell'indebitamento gli interessi rispetto a quei fondi. Il fatto che si stia prendendo questa decisione, legittima, che noi non avevamo preso perché non la condividiamo, non significa che si sta calando all'interno dei conti dei conti dello Stato necessariamente quello che era stato detto dell'EUROSTAT, ma si sta facendo questa operazione perché è stato reputato necessario scaricare il bilancio delle Ferrovie dello Stato per i *bond* che le Ferrovie dello Stato devono devono emettere. Tutto un ragionamento di contabilità che invece, rispetto alla denunzia fatta dal senatore Legnini, ha soltanto delle connotazioni di falsità. Tre: non non ci si può venire a dire che loro hanno aumentato i fondi per l'ANAS e per le Ferrovie dello Stato, perché il conto che dev'essere fatto sul 2007 (che è poi quello che in parte si fa, ma che si cerca di

riconsiderato le cifre con le manovrine di primavera. Il conteggio dev'essere fatto quindi non sulle cifre impostate in bilancio, ma sulle effettive spese. tutto quello che c'è nel Paese è evidente, la quantità di cantieri aperti, di opere definite; il consenso che abbiamo tuttora e che abbiamo avuto per le iniziative che, dal punto di vista infrastrutturale, sono state prese dal Governo Berlusconi è evidente. È evidente ancora che la falsità dei discorsi fatti dai colleghi della maggioranza finisce per dispiacerci, perché significa dare una comunicazione al Paese che è la negazione di quello che la democrazia dovrebbe fare, cioè un onesto confronto: ma di onesto in quest'Aula, da stamattina, non c'è nulla. C'è soltanto una deprecabile comica che rappresenta il disdoro delle istituzioni e che ancora una volta mi dà dovere di appellarmi alla Presidenza del Senato perché quello che ci è stato annunciato, cioè la fine di questa commedia, sia compiuta e che finalmente si abbia il testo del maxiemendamento della finanziaria perché è questo che tutti stiamo aspettando. Non discorsi inutili, quindi, ma serietà, augusti colleghi della maggioranza!

Il collega Legnini nelle sue valutazioni ha detto cose contabilmente esatte, tecnicamente sbagliate, politicamente mistificatorie. Infatti, nel precedente intervento del collega Albonetti è trapelato un problema interno alla maggioranza

secondo il manuale Cencelli di questo Governo e di questa maggioranza la sua parte politica ha avuto un peso più istituzionale e meno ministeriale, ha in qualche modo sollevato l'argomento, con grande pacatezza e prudenza. Ma vedete, signor Presidente e onorevoli colleghi, le parole del senatore Legnini sono gravissime, perché sono la prova di quanto da noi sostenuto ieri, nella richiesta di sospensiva, a proposito di questo bilancio: esse sono la prova che questo bilancio è falso, contiene dei numeri falsi e contiene dei numeri che dipenderanno da un maxiemendamento che a questo punto nessuno conosce. Il Senato sta approvando tabelle e numeri che sono palesemente smentiti da ciò che dice il Governo. Il senatore Legnini ha infatti affermato che le maggiori entrate del 2006, nel 2006 sono state utilizzate per coprire due sopravvenienze passive e cioè la sentenza sull'IVA, per circa 13 o 14 miliardi, e lo spostamento del debito dall'ISPA allo Stato per circa 13 miliardi. Non a caso questa somma è pari a 25 miliardi, perché il di più di entrate nell'anno 2006 - dichiarato formalmente dal vice ministro Visco in Commissione: atto formale consegnato

Con queste maggiori entrate nel 2006, ha appena detto il collega Legnini, il Governo ha coperto due sopravvenienze passive. Ovviamente non ha tenuto conto che sono due voci di debito pregresso che non hanno niente a che vedere con l'indebitamento netto di competenza dell'anno 2006, che è un concetto di flusso e non di *stock*. Ma lasciamo perdere questa tecnicalità. Quindi, l'indebitamento netto di competenza dell'anno 2006, stimato al 3,6 per cento del PIL, non balza perché ci sono due poste di debito pregresso. Aumenta il debito pubblico che emerge, ma non c'entra niente con il flusso di indebitamento: è la solita confusione ragionieristica tra conto economico e stato patrimoniale. Mi sono sentito dire questa mattina in una pubblica trasmissione da un Vice ministro di questo Governo che il TFR dei lavoratori presso le imprese non è mai stato registrato a debito, quindi mi rendo conto che c'è un po' di confusione nella maggioranza di fra Luca Pacioli. Ma, collega Legnini, se è vero quello che ha appena detto, che ne è di queste entrate pubbliche nel 2007, visto che il Governo ha ribadito che per il 2007 di questi 38 miliardi in più di entrate 2006 ne considera strutturali e permanenti (e li ha contabilizzati in queste tabelle che stiamo discutendo ed approvando) solo 5 miliardi, quando la tabella del Ministero dell'economia indica che strutturali e permanenti sono almeno 25-28 miliardi? Questo è il dato di falsità per il quale abbiamo chiesto ieri la sospensiva. In altri casi, nella precedente legislatura, con altro Presidente della Repubblica, questa tabella non sarebbe mai passata. Vengo ora alla tabella specifica del Ministero delle infrastrutture: perché votiamo contro? Perché rispetto alla falsità complessiva del bilancio di previsione dello Stato,

(è quello che ha appena detto il collega Legnini): sono previsti investimenti infrastrutturali, ma questo noi non lo sappiamo dire e non lo possiamo dire, perché sono previsti 6 miliardi di investimenti infrastrutturali finanziati con un'appropriazione indebita, cioè spostando il TFR dei lavoratori dalle imprese all'INPS.

quale sarà la decisione dei lavoratori, se opteranno per spostare il TFR nei fondi pensione o lo lasceranno nelle imprese, alla mercé delle grinfie di questo Governo, che l'inoptato glielo sposterà, senza nessuna formale dichiarazione scritta del lavoratore? Infatti, delle due, l'una: o i lavoratori, entro luglio dell'anno prossimo, opteranno per spostare tutto il TFR ai fondi pensione, e allora questa tabella dovrà avere zero

contravvenendo alla legge, perché il TFR è salario differito e nella motivazione contabile dell'ISTAT si afferma che è considerabile come un di più di contributi sociali, altra falsità statistica nella falsità sostanziale.

tutto il TFR ai fondi pensione, che numero ci ritroveremo a luglio, su questa tabella, visto che scatterà automaticamente il fondo negativo che azzera i 6 miliardi?

lasciandolo nelle imprese, lo spostamento all'INPS sarà - ripeto - un'appropriazione indebita, ma sarà comunque una copertura a debito delle infrastrutture, non coperta. E allora mi domando: questi 25 miliardi di entrate in più nel 2006 che avete usato per coprire i due debiti dell'IVA e dell'ISPA, che ci sono strutturalmente nel 2007 (lo dimostra la tabella del Governo), perché non avete voluto metterli nei numeri del bilancio preventivo e con questi finanziare sul serio le infrastrutture, con le tasse che pagano i cittadini italiani, non con un'appropriazione indebita, una tecnicalità formale e con la quale comunque sono finanziate a debito?

euro non riportate nel bilancio del 2006. Voi operate un altro trucco contabile, scaricando sul 2006 i 12.700 milioni di euro delle Ferrovie dello Stato

periodo in cui voi siete stati al potere, è stata programmata una sola, unica opera infrastrutturale importante: l'alta velocità da Roma a Napoli. Per il resto, è stato il deserto assoluto. Perché oggi possiamo parlare di centinaia di cantieri aperti? Per un motivo molto semplice: è stato dato al Paese, al Governo, al Parlamento lo strumento per poterlo fare,

È che voi avete fermato tutto: avete fermato il MOSE e fermate, attraverso i governatori a voi vicini, i gassificatori che sono importantissimi per la politica energetica del Paese.

Neanche uno, e non soltanto perché sono mutate le condizioni climatiche, ma perché è l'unico *hub* italiano dotato di strutture elettroniche per cui gli aeroplani possono atterrare in ogni caso. Ho detto questo a

onorevoli senatori, ieri, in un dibattito molto interessante - almeno tale lo reputo dal punto di vista politico è stato un impegno da parte del presidente Marini di sollecitare almeno per le ore 12 la presentazione del maxiemendamento. Poiché i colleghi senatori

Vista la cortesia che il Ministro ha usato, almeno questa volta, nell'informarci, ho ritenuto di dire al Ministro che il Gruppo di Alleanza Nazionale

un fallimento da parte della politica di questo Governo. Siamo, quindi, di fronte ad un dibattito politico molto interessante anche da questo punto di vista e il maxiemendamento ci chiarirà se il Governo ha cercato di rimediare a questo fallimento della politica, sostenuto dall'onorevole Fassino. Ci sarà un ampio dibattito e in questi giorni il Senato sarà veramente protagonista della vita politica italiana.

relativa all'andamento dei nostri lavori e alla presentazione del maxiemendamento da parte del Governo, sarà il presidente Marini, che sta venendo in Aula, ad informare l'Assemblea sull'andamento di questa vicenda.

ha fatto un intervento a metà tra dichiarazione di voto e intervento nel quale sostanzialmente, pur riconoscendo la legittimità degli interventi che alcuni colleghi stavano facendo in dichiarazione di voto

nella presentazione del maxiemendamento da parte del Governo, evitiamo di trascinare la votazione sul bilancio in maniera

anch'io. Vorrei ritornare un attimo alla discussione di ieri, quando, ad un certo punto, è stato posto il problema di passare - giustamente, secondo me - al voto del disegno di legge di bilancio. Ieri mattina - ho rivisto il testo stenografico - ero stato abbastanza preciso. Certo, i Capigruppo dell'opposizione avevano con forza posto il problema della necessità di un dibattito forte sulla finanziaria, con i tempi necessari. Però si era trovato un punto di equilibrio tendente ad avviare il dibattito, come poi è avvenuto ieri, concentrandoci più sugli

solo ricordarle, Presidente, che quando avviene il deposito del maxiemendamento è prassi, secondo le innovazioni introdotte dal presidente Pera,

Volevo anche stigmatizzare il fatto che l'invito che lei ha rivolto all'Aula, e che noi abbiamo promosso, era indirizzato alla maggioranza perché, fino ad oggi, il mancato rispetto dell'impegno di ieri non era stato colpa nostra ma dolo della maggioranza.

perché il mio intervento, come altri senatori, lo svolgerò nell'ambito della discussione sul maxiemendamento. Volevo soltanto che restasse a verbale che stavo per fare, prima di questa discussione correttamente procedurale,

le cose sostenute dal senatore Legnini in ordine ai conti in disordine di ANAS, Ferrovie, ISPA ed alta velocità sono purtroppo assolutamente vere e con questo provvedimento, nell'ambito sia del bilancio che della legge finanziaria, tentiamo di porre rimedio e di dare una prospettiva a questo problema.

perché in questa finanziaria, pur avendo una quantità di risorse rilevante, avete tagliato le poche risorse che pure erano state stanziate sulla Genova-Milano e sulla Milano-Verona, che rientrava nella programmazione

mi voglio astenere perché non è possibile passare sotto silenzio un intervento dai contenuti falsi e propagandistici come quello del senatore Legnini: falsi perché gli atti prodotti da questo stesso Governo lo smentiscono. Faccio riferimento alla ricognizione del CIPE del mese di settembre per confermare quanto asserito dal presidente Grillo: fatte cioè cioè 100 le opere programmate dal Governo Berlusconi, 30 sono interamente finanziate, 50 parzialmente finanziate e 20 soltanto vedono ancora nella fase di progettazione il loro *iter* procedurale. Ed il complesso dei finanziamenti supera i 50 miliardi di euro. Questo non lo dico io, ma il Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalla vostra maggioranza a luglio e lo dice l'atto ricognitivo del CIPE al 30 settembre di quest'anno. Ciò premesso, approfitto del tempo restante per una denuncia: abbiamo fatto una programmazione che ha trovato il suo momento di unità all'interno del piano Van Miert che conteneva tre corridoi fondamentali nel nostro Paese: il corridoio Genova-Rotterdam, il Corridoio 5 ed il corridoio Berlino-Palermo, che enfatizzava la Piastra logistica della Sicilia. Con l'eliminazione del corridoio tirrenico e del ponte sullo Stretto, il corridoio Messina-Palermo è morto; con la valutazione di impatto ambientale da effettuare sul progetto definitivo, invece di accettare quella già fatta sul Frejus, è morto anche il Corridoio 5. Questo sarà un problema della prossima legislatura perché i tempi per la valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo si misurano in alcuni anni. Di più, con la morte del terzo valico è morto anche il corridoio Genova-Rotterdam. Ebbene, abbiamo impiegato cinque anni per costruire una pianificazione che puntasse allo sviluppo del Paese. A voi sono bastati sei mesi per smontare tutto, senza sostituirlo con altri strumenti di pianificazione! E poi vi meravigliate se il 2 dicembre milioni di persone manifestano contro questo Governo!

le infrastrutture del nostro Paese, in modo particolare il Corridoio 5. Oggi due quotidiani importantissimi hanno evidenziato che la Francia sta già costruendo 300 chilometri di linee in alternativa il nostro Paese corre veramente il rischio di essere bypassato e riportato verso le economie del Sud del Mediterraneo. Si tratta di una circostanza molto pericolosa.

che ritengo molto grave ed estremamente puntuale per la discussione che stiamo svolgendo su questa finanziaria. La Standard & Poor's si riferisce alla manovra di bilancio del Governo Prodi

con una riduzione solo marginale del *deficit*, ottenuta per lo più con aumenti fiscali e non con riduzioni di spesa, accompagnata da incertezza sulle entrate, dalla lotta all'evasione e dal carattere debitorio del trasferimento del TFR. Questa è una puntuale bocciatura della finanziaria del Governo Prodi e noi dovremmo avere la coscienza civica e politica di farne tesoro.

Il debito che abbiamo consegnato, pertanto, era quello effettivamente e anzi era esaltato dal fatto che l'intero debito e gli interi fabbisogni erano già stati scontati. Questa è una mera postazione di tipo contabile che consente alle Ferrovie di cancellare i loro debiti. per chiarire che l'aumento dell'indebitamento netto è soltanto una questione che assume un rilievo tecnico, ma che gli effetti sostanziali erano stati correttamente scontati nel nostro debito. Ciò che abbiamo lasciato a questo Governo è stato il pagamento di tutto ciò che era

del fatto che stiamo approvando una tabella che può essere modificata da qui a poche ore dal maxiemendamento, visto che il Governo stesso ha detto che spera che nel maxiemendamento ci siano risorse in più per il tema generale della sicurezza. Sottolineo ancora una volta l'assoluta disinformazione non solo dell'opposizione, ma anche della maggioranza rispetto ai numeri veri che state approvando in questo momento. Il Governo non ha risposto ancora alle questioni poste dal senatore Cossiga. Si tratta di questioni importantissime e gravissime in base alle dichiarazioni del senatore Cossiga, ma sta di fatto che il Governo non ha risposto ancora a se stesso, perché tutte le questioni che stiamo ponendo, sin da ieri e prima in Commissione, relativamente al bilancio di previsione per l'anno 2007, non hanno ricevuto risposta. Il Governo non ha risposto a se stesso perché con i dati che ha reso ufficiali e ha reso alle Camere avrebbe dovuto fare l'assestamento e dice che non lo fa; non risponde a se stesso; non risponde alla sua maggioranza che palesemente non ha la più pallida idea di che cosa verrà inserito nell'emendamento; non risponde al senatore Cossiga. Francamente, vorrei sapere a chi risponde questo Governo quando scrive e decide nel segreto delle sue stanze la finanziaria e la destinazione delle tasse degli italiani. Capisco che la maggioranza sia un po' in fibrillazione, perché una cosa l'ha capita che ci sono 25 miliardi in più di entrate dovute all'andamento del 2006, che con la finanziaria porteranno a casa altri 35 miliardi di entrate e che questi soldi degli italiani

di portare a casa queste risorse per poi gestirle a loro discrezione e per farci essere tutti più sudditi e meno liberi cittadini. Per questo votiamo contro l'articolo 12, ma chiediamo alla maggioranza o a chi vota a favore se è consapevole di che cosa sta votando e se è sicuro che i numeri scritti nella tabella 12 fra un'ora e mezza o due ore e mezza non verranno modificati dal maxiemendamento che presenterà il Governo. Allora, che cosa avremmo votato questa mattina, signor Presidente? Ecco dove il Governo non risponde a se stesso, oltre che non rispondere ancora al senatore Cossiga; doppia non risposta, in questo caso.

ci riferiamo a due capitoli di spesa del bilancio del Ministero della salute; sono molto importanti per noi e vorremmo che almeno si ripristinasse il quantitativo di finanziamento previsto nella passata legislatura, dato che c'è stato un decurtamento in questa. 15.Tab.15.2 parla del sistema informativo sui trapianti. Sappiamo quanto è importante il dono di organi

Anche su questo capitolo chiediamo almeno di ripristinare i finanziamenti predetti e spero che la collega Rita Levi Montalcini, che è donna di grande ricerca, appoggi il nostro emendamento. *(Applausi

ovviamente contrario. È del tutto evidente, infatti, che, essendo in sede di bilancio, non è facile modificare l'equilibrio di tabelle, se non c'è un quadro generale, visto un impegno a tagliare tutto. Per altro in finanziaria vi sono emendamenti nel merito che affrontano tale questione.

ma almeno ci si risparmi l'offesa di dire che «ovviamente» gli emendamenti vengono respinti.

Presidente, le questioni poste dalla senatrice Bianconi sono molto importanti, talmente importanti che negli interventi previsti dalla legge finanziaria

Signor Presidente, trattandosi di materia di Ministero dell'università

quella che mi permetto di sottoporre al Governo, da cui desidererei una risposta. Giunge notizia che il maxiemendamento alla legge finanziaria sia composto di ben 1.400 commi, che è un *record* assoluto nella storia della Repubblica, una quantità così esondante di norme ovviamente non serve ad altro che a creare un sistema di potere e di regali. Cantoni ha detto che c'è un *downgrading* del *rating*: probabilmente dipende anche dal fatto che le aziende e le società di *rating* hanno iniziato a considerare cosa può essere veramente il testo di questa finanziaria.

sotto la soglia psicologica dei mille.

che le università dovranno pagare, si prevede un aumento di circa 350-400 milioni di euro. Dunque, il rischio è che i docenti universitari, il personale dell'università non potrà vedersi liquidate queste somme. Voglio anche replicare a quanto detto poco fa

nella Nota di variazione al bilancio, infatti, si parla di una cifra che passa da 42 miliardi 249,9 milioni a 42 miliardi 170 milioni, senza tener conto, per altro,

devo anche aggiungere che non c'è alcun recupero del pesante taglio effettuato dalla legge Bersani sul settore università, pari a circa 250 milioni di euro. La legge Bersani, per altro, un taglio l'aveva fatto anche sul settore dell'istruzione.

Su di lui, sulla sua richiesta di essere accompagnato oltre la vita in piena consapevolezza, si esprimeranno quelli che sono gli attuali decisori: gli esperti del Consiglio superiore di sanità

Su di lui i medici esporranno - come hanno fatto in questi giorni - i dilemmi e le obbligazioni del loro codice deontologico. Non è di questo di cui oggi voglio parlare. Ognuno di noi sulla linea di confine che passa tra l'accanimento terapeutico e l'eutanasia l'eutanasia ha opinioni, dubbi oppure certezze. Comunque ognuno di noi avrà come legislatore propositi e determinazioni. Oggi voglio solo rivolgere un pensiero a Welby che, come punta di un *iceberg* di un mondo più vasto di persone sofferenti, chiede attenzione, ascolto e dignità.

hanno espresso la propria disponibilità per sabato sera per testimoniare e dare un segnale di attenzione a questa richiesta di dignità. 130 nostri colleghi hanno detto che in qualche modo saranno accanto alla sofferenza di Welby. Desidero solo lasciare testimonianze in quest'Aula che la concitazione di questi giorni non ci ha resi insensibili, né ciechi, né indifferenti, di fronte a questa stoica e straziata battaglia. Ha scritto Barbara Spinelli domenica scorsa su «La Stampa»: «Il volto di Piero Welby che da tempo ci accompagna con il suo sguardo, non è un volto pacificato, passivo, docile. E' un volto molto severo che interroga, un volto d'intranquillità che esige da ciascuno di noi pensiero profondo». Non ho voluto né sono in grado di lasciare un pensiero profondo. Desidero solo lasciare traccia in questa Aula di un pensiero di gratitudine, di omaggio all'uomo Piergiorgio Welby, e di profondo e quasi intimidito rispetto; ma anche un pensiero di speranza. La speranza che in questi giorni che corrono e che si stanno per lui consumando - come dice il professore Umberto Veronesi - la sua battaglia non sia vana. *(Applausi dai

poche parole per associarmi a quanto detto dalla collega Negri. Ho già dato la mia adesione alla veglia di sabato prossimo

che Piergiorgio Welby propone al Paese e alla politica. La propone con coraggio, con determinazione e con estrema consapevolezza,

quindi non ideologica né teologica. Una richiesta che viene dall'intelligenza delle cose, dall'intelligenza di sé, dall'intelligenza dei rapporti e dall'intelligenza rispetto a quanto la scienza ha fatto e a quanto non è ancora in grado di fare. Proprio per questo assume su di sé e rivendica di assumere sulla responsabilità di ciascuno la scelta di come concludere la propria vita in una condizione nella quale non è dato al singolo decidere se vivere

Presidente, accolgo il suo invito alla brevità e mi limiterò ad esprimere la mia adesione alle considerazioni svolte dalla collega Negri e a testimoniare anch'io la solidarietà verso la battaglia intelligente,

il suo atteggiamento merita rispetto e solidarietà da tutti noi.

è effettivamente una situazione di accanimento terapeutico che non ha nulla a che vedere con la discussione in corso nella Commissione igiene e sanità del Senato circa possibilità di pervenire ad una legge sulle direttive anticipate di trattamento. Mi sembra superfluo sottolineare che le direttive anticipate di trattamento un disegno legislativo che riguarda chi non può più esprimere la propria opinione e decisione rispetto alle terapie. ci troviamo in una situazione in cui il consenso informato, che rappresenta un fatto civile e obbligatorio, rispetto ad una terapia (qualunque essa sia) può essere espresso dal paziente. Credo che di questo fatto dobbiamo tutti

che tanto ha commosso tanta parte della nostra pubblica opinione. Vorrei, però, riprendere anche quanto poc'anzi affermato dal senatore Marino: ciò che viene presentato alla pubblica opinione è un caso in cui si afferma esistere un accanimento terapeutico. Non so se ciò sia vero o falso (possono giudicarlo soltanto i medici che ne hanno cura), ma, certamente, è in contraddizione stridente con il tentativo di fare della sofferenza di Piergiorgio Welby un modo per premere sulla pubblica opinione al fine di ottenere l'approvazione di una legge sull'eutanasia. Credo che questo sia irrispettoso, per la condizione dell'essere umano concreto che soffre, oltre che indebito, per quel che riguarda la correttezza del dibattito politico; ritengo, infatti, che abbia immiserito anche la partecipazione che tutti noi sentiamo,